senza «no no», da una parte, o «sì, sì», dall'altra. A questo riguardo vorrei ricordare, soprattutto ai colleghi senatori che non sono Presidenti di Gruppo, che stiamo ancora lavorando nell'ambito di una decisione assunta dai Gruppi all'unanimità che riguarda

quando è toccato a me presiedere la seduta ho sentito qualche sollecitazione di troppo, che ovviamente devo rispettare e far rispettare il Regolamento, che prevede che sul processo verbale si possa intervenire così come sull'ordine dei lavori,

Non è un fatto formale. Ieri sera abbiamo rischiato un *vulnus* all'interno di quest'Aula. Voglio vedere questa mattina se recuperiamo, ma non posso non tener conto di cosa è accaduto nelle precedenti votazioni, quando vi è stato il voto di fiducia. Ho preso a caso questa mattina

favorevoli 160; contrari 1. La somma è sempre 161. Il Presidente non è conteggiato mai.

Signor Presidente, mi associo alla richiesta del collega Matteoli. Rifacendomi alle sue preventive dichiarazioni,

sovrana; libera di parlare sull'ordine dei lavori, laddove ve ne siano motivazioni legittime. Non credo e non ritengo che spetti e rientri nei compiti della Presidenza strozzare un dibattito. Se la sua intenzione è questa, lo dica subito. Ci auguriamo che così non sia perché il *vulnus* di ieri sera è ancora caldo per poter accettare serenamente la sua preventiva dichiarazione di voler porre ad un certo momento della giornata lo stop agli interventi. Mi auguro che questo non avvenga, al fine di non indurci a manifestazioni di contestazione ancora più gravi rispetto a quelle di ieri sera. Il dato politico di ieri sera è sotto gli occhi di tutti e la stampa di oggi lo testimonia, e lo sarà ancora di più nella giornata odierna perché è evidente che faremo sentire la nostra voce. Ieri sera il *quorum* sulla fiducia al Governo Prodi non c'era. È stato raggiunto grazie al computo della ipotetica presenza alle votazioni - presenza che non vi era stata - del Presidente del Senato.

È eccessivamente sintetico; non contiene l'esatta scalettatura dei lavori. Il Presidente del Senato, quando ha letto

presenti 160; votanti 159; maggioranza 159. Questo non ha fatto. E noi ci chiediamo per quale motivo. Non vogliamo Non vogliamo pensare che questa omissione sia stata realizzata proprio per nascondere una anomalia che sarebbe saltata in maniera evidente agli occhi di tutti. Noi per fortuna ce ne siamo resi conto, abbiamo subito denunziato in Aula questo stato di cose e da lì è venuta fuori la verità, una verità che abbiamo contestato e che non abbiamo riscontrato nel processo verbale della seduta di ieri sera, è un verbale che non condividiamo e che non approviamo,

Presidente, gli autorevoli Presidenti dei Gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia hanno ripreso, per chiedere la verifica del numero legale, il tema che abbiamo affrontato ieri sera in Assemblea e che ha visto accendersi un dibattito non tanto sull'interpretazione del Regolamento, che è chiara, non tanto sulla prassi del Senato, che è altrettanto chiara, quanto sulla situazione che si è venuta a determinare a seguito della lettura dei risultati. avevo già previsto, ieri sera, nel mio intervento, e vedo che è riportato correttamente nel verbale, che il presidente Matteoli e il presidente Schifani, ripeto ancora questa mattina, in buona fede, presi dalla circostanza e dalla concitazione, avrebbero tratto un'impressione sbagliata rispetto alla verità dei fatti. Prendo atto, questa mattina, che il giudizio non è più sulla legittimità dei nostri comportamenti, ma è un giudizio politico sulla situazione che viviamo e cioè che

la questione in un alveo che è molto più consono al dibattito che dobbiamo svolgere, perché onestamente devo dire, se mi è consentita una battuta polemica, che ieri sera c'è stata una caduta di stile, perché mettere la Presidenza dell'Assemblea in una condizione come quella di ieri sera, per chiunque fosse stato al banco della Presidenza, magari anche un collega

che un minimo di riflessione sulla questione debba intervenire e quindi non tanto sul processo verbale, perché condivido anche il suo indirizzo di non approfittare in maniera impropria dell'argomento all'ordine del giorno per porre problemi d'interpretazione delle norme del Regolamento e, se mi consentono i colleghi dell'opposizione, di comprensione anche della nostra Costituzione. Se i colleghi leggessero bene l'articolo 64 della Costituzione troverebbero le risposte a tutte le loro argomentazioni. Così come, il presidente Matteoli, che ho visto questa mattina essere ancora più responsabile di ieri sera, ha giustamente letto quello che è accaduto, ma se lo leggesse con serenità, si accorgerebbe che il Presidente dell'Assemblea ha parlato, appunto, di votanti e non di presenti, per cui ha riferito all'Aula qual era la situazione dei votanti e l'ha riferita correttamente.

i segretari, che hanno il compito di coadiuvare il Presidente nell'individuazione dei votanti, firmano un verbale e sono loro che nella firma del verbale certificano il numero dei presenti, oltre a quello dei votanti. Come, appunto, prevede la nostra Costituzione, bisogna verificare prima il numero dei presenti e poi il numero dei votanti. Signor Presidente,

se necessario, facciamolo anche in Aula, perché è un tema che riguarda tutti. Ovviamente, non è questa la sede, dovremmo aggiungere questo punto all'ordine del giorno, dovremmo parlare solo di questo e non mi pare che sia l'argomento più rilevante ai fini del buon andamento dei nostri lavori. Tuttavia, aggiungerei alla riflessione che invito il Presidente del Senato a fare, nell'occasione che riterrà, due questioni che cito soltanto senza trattare. In primo luogo, tra

Presidente, è in possesso di un verbale della votazione che è stato firmato, firmato- ripeto - da due segretari che hanno assolto compiutamente il loro dovere.

che, materialmente, firma il verbale della seduta. Non è proprio immaginabile che si possa considerare assente il firmatario del verbale della seduta. Signor Presidente,secondo la legge comunale e provinciale per chiedere la verifica del numero legale basta un solo consigliere. Quel consigliere viene computato ai fini della presenza. Non può essere diversamente. Chi esercita una funzione istituzionale, nel momento in cui la esercita, non può essere

i richiedenti della verifica del numero legale, ancorché non premessero il pulsante, dovrebbero essere considerati assenti? Ma è mai possibile che il richiedente della verifica del numero legale possa essere considerato assente? Sono questioni che esistono.

C'è un'altra questione, che vorrei che fosse esaminata e anche questa la cito soltanto. È la questione, da sempre posta e mai risolta anche qui al Senato, tra assenza nel voto, astensione nel voto e assenza o astensione dal voto. Se lei, signor Presidente, affronta questo argomento, vedrà che c'è materia di discussione. Riconosco che i presidenti Matteoli e Schifani hanno ragione: c'è materia di discussione. In questi casi, signor Presidente, il nostro Regolamento - e devo dire la verità anche quello della Camera - è molto carente, perché non distingue tra assenza nel voto e assenza dal voto. Il presidente Casini come il presidente Violante hanno risolto tale questione ritenendo che fosse presente colui il quale è lì e si vede. Signor Presidente,credo si debba accogliere la richiesta di una riflessione. Prendo atto che rispetto a ieri sera c'è un diverso stile nel porgere il problema e anche io mi associo alla necessità che, nei modi e nelle forme che la Presidenza riterrà opportune, si possa affrontare questo argomento.

poiché siamo all'inizio di una lunga due giorni di lavoro parlamentare, vorrei rivolgermi brevemente ai colleghi Matteoli e Schifani che sono stati protagonisti del dibattito sollevato ieri sera nello scorcio finale della seduta e questa mattina sono tornati a parlare sul verbale. Proprio per il verbale vorrei che rimanesse la nostra valutazione sulle questioni regolamentari che essi hanno posto.

intervenire anche sul significato politico delle questioni che lei ha sollevato ieri sera e che siete tornati a ribadire questa mattina, perché credo che su questo aspetto, che è politico, del nostro confronto noi dobbiamo cominciare a parlarci con franchezza e a dire ciascuno quale è il proprio giudizio e anche quali sono i propri proponimenti per il futuro. Allora, per quanto riguarda la questione regolamentare, è giusto promuovere l'approfondimento che chiedeva prima il collega Boccia. Tuttavia, voglio dire, affinché rimanga anche nel verbale della seduta di questa mattina, che in ciascuno dei nostri voti la presenza del Presidente del Senato, di colui che presiede l'Assemblea, è implicita, è un presupposto, è innegabile e ogni volta è registrata. La macchina che regola questa registrazione delle nostre presenze è disposta in modo tale da calcolare sempre e, quindi, da presupporre la presenza in Aula, ai nostri lavori, e quindi anche al voto, del Presidente del Senato.

deve partire da questo dato di cui ieri sera non sembravano pienamente consapevoli molti degli intervenuti. Altra questione, collega Matteoli, è quella politica da voi sollevata ieri sera e che continuate e continuerete, è un vostro diritto, a sollevare nel dibattito pubblico. Il numero legale ieri sera è stato raggiunto per una sola unità. La maggioranza che si è espressa attraverso il voto di fiducia aveva ieri sera un margine certamente ristretto e la vostra battaglia di opposizione

con l'*handicap* per noi che il margine di maggioranza del centro-destra, sulla base di una diversa legge elettorale, era molto più ampio. Quindi, nessuno vuole contestare la legittimità dei giudizi politici che formulate, ma io esprimo una preoccupazione che dal giudizio politico, dalla polemica politica che si sviluppa in questa Aula e fuori, che credo sia utile alla vita democratica del Paese, si passi a contestare un'applicazione pacifica del Regolamento e poi, secondo un copione che ho visto più volte riproporsi in questi giorni, a un attacco diretto contro il Presidente del Senato. Noi abbiamo polemizzato con il presidente Pera nella scorsa legislatura per le posizioni che assumeva, per i giudizi che esprimeva, ma sempre, collega Matteoli, con una sorta di *stop* *and* *go*, per cui ci fermavamo di fronte alla carica e alla funzione del Presidente del Senato. Voi dovreste - ma non mi permetto di dare consigli all'opposizione - essere consapevoli della necessità di non spostare la lotta e la battaglia politica - che deve essere rivolta contro di noi e contro il Governo - verso le istituzioni che reggono questa Assemblea,

però, senatore Boccia, quando c'è un dubbio legittimo sull'atto più alto di una democrazia, cioè quello del voto, abbiamo il dovere di acclarare fino in fondo cosa è accaduto, in modo che ciò non costituisca precedente e in modo che poi i nostri lavori si sviluppino attraverso un dibattito, anche duro ma con argomenti politici. Gradirei che l'occasione di ieri sera ci facesse in maniera definitiva capire

se questa infatti è stata la sua impressione vuol dire che qualcosa nelle mie parole non è andato per il verso giusto. Volevo dire precisamente il contrario, come mi pare del resto, senatore Schifani, di aver dimostrato ieri mattina quando non ho assolutamente impedito un dibattito che ritengo sempre legittimo, ovviamente nelle forme dovute, non nelle forme estreme che ieri mattina esso ha assunto e che mi auguro non assuma più. Ho fatto, mi pare non esorbitando dalle mie responsabilità, riferimento al programma di lavoro che abbiamo, che - come lei sa meglio di me per antica esperienza è un programma impegnativo a cui guarda anche la società italiana nel suo complesso. Quindi, ovviamente non c'è da parte mia nessuna volontà di strozzare il dibattito, del resto anche questo primo accenno di discussione lo dimostra. C'è un principio di ragionevolezza che io, ad un certo punto, ovviamente insieme a voi, dovrò far pesare per quanto riguarda

C'è un problema di tessera, risolvetelo, per cortesia.

chiusa la votazione

Per favore, se non si può lo decide la Presidenza, fino a prova contraria. STORACE *(AN)*. Signor Presidente, prima ho ascoltato un appassionato intervento del senatore Brutti che spero sia nelle condizioni di ascoltare - a tutela dell'istituzione Presidenza del Senato; egli ha detto che non si può attaccare il Presidente del Senato.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, la votazione di fiducia dell'odierna seduta... *(Brusìo)*. PRESIDENTE. Senatore Barbato, aspetti un attimo il deflusso.

Colleghe e colleghi, la votazione di fiducia dell'odierna seduta ha per oggetto un provvedimento che esprime la chiara volontà dell'Italia di ribadire con forza le proprie responsabilità di Paese impegnato nella politica internazionale. È un voto che riguarda la partecipazione a ben 24 missioni, nelle quali la nostra Nazione ha da sempre apportato l'impegno massimo e il suo prezioso contributo, al fine di raggiungere il sacrosanto obiettivo della stabilizzazione dei conflitti che mettono in ginocchio tante parti del mondo; tale obiettivo deve rimanere scopo comune delle massime potenze. Altro scopo delle missioni in questione è quello di ottenere il rafforzamento dei processi democratici in Paesi che hanno da poco intrapreso questo lungo percorso. Queste sono le motivazioni che spingono i Popolari-Udeur a votare con convinzione nel merito del provvedimento, esprimendo un voto positivo di fiducia su di esso. Voteremo per le missioni in Iraq e in Afghanistan, ma anche per le altre importanti missioni di supporto in Paesi come Bosnia, Kosovo, Albania, Eritrea, Macedonia, i quali, dopo avere subito anni di devastazioni e sofferenze, sicuri e forti dell'appoggio internazionale, tentano di ricostruire il proprio futuro. Non votare questo provvedimento significherebbe, quindi, assumere un atteggiamento di indifferenza assolutamente condannabile poiché - lo ribadisco - l'Italia ha delle precise responsabilità internazionali, cui non può sottrarsi, derivanti non solo dalla sua posizione politica ed economica, ma anche dell'impegno umanitario e di solidarietà assunto. Per quanto attiene alla missione "Antica Babilonia" in Iraq, il rientro del contingente militare di stanza nella regione di Dhi Qarcorrisponde ad un preciso mandato elettorale che questa maggioranza intende puntualmente rispettare. Occorre necessariamente finanziare tale rientro che dovrà svolgersi in maniera ordinata e concordata con i nostri alleati e con il Governo iracheno legittimamente insediato. Si tratta di mettere in atto la cosiddetta *exit strategy* che, come qualcuno degli esponenti di Rifondazione Comunista ha avuto modo intelligentemente di sottolineare, deve costruirsi con pazienza, senza forzature controproducenti. Queste forzature - aggiungo io - finirebbero solo per indebolire la coalizione di Governo e a fare perdere credibilità all'Italia nel contesto internazionale. Lasciatemi spendere qualche parola di encomio per quanti hanno partecipato in maniera esemplare, apportando il loro preziosissimo contributo ad una missione che dura da oltre tre anni. Mi riferisco ai tanti giovani che hanno affrontato con coraggio le insidie e i pericoli di una terra straziata dal conflitto, talvolta a costo della propria vita, per rispondere al compito di garantire la sicurezza dei più deboli fra gli A loro va un accorato e - spero - concordato grazie. Passando poi alla tanto dibattuta questione della missione in Afghanistan, questa - com'è noto - nasce sotto l'egida delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 1368 che ha legittimato la NATO a porre in essere operazioni - anche con il ricorso all'uso della forza - utili al ripristino della democrazia e al contrasto del terrorismo internazionale. In tale cornice opera il contingente italiano a partire dal 2002 con l'ISAF.

Cosa diversa è l'operazione *Enduring Freedom* che nasce da un accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti per il quale il nostro Stato si limita a fornire solo due unità della Marina militare per il pattugliamento di alcune zone di mare fuori dal territorio. Certamente la situazione di quelle zone si sta rivelando ancora estremamente critica e per questa ragione ci è stato rivolto un appello dal segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan al rafforzamento della nostra presenza, appello che accoglieremo e al quale non potremo sottrarci. Pertanto con la votazione odierna, confermeremo il nostro contributo materiale a sostegno della missione in quei territori e contestualmente ci impegneremo a fornire un apporto prezioso nel dialogo internazionale con l'obiettivo comune di ricercare la soluzione più adatta a fronteggiare le crisi democratiche dell'Afghanistan. A tale proposito mi piace concludere riportando una frase assai significativa di un editoriale del quotidiano «Avvenire»: «Quando la forza e il diritto procedono insieme, nella condivisione della responsabilità

automaticamente impone un vincolo alla nostra sovranità nelle modalità di scelta. Ogni volta che si aderisce ad un organismo collettivo, si accetta poi di fare parte di quell'organismo rispettandone le decisioni e gli orientamenti. gli orientamenti. Ciò è avvenuto e credo che questa sia la questione vera, anche nei confronti di coloro che, con qualche difficoltà, votano questo provvedimento. Stare in un organismo internazionale significa accettarne le regole e le risoluzioni, contribuendo sì ad adottare risoluzioni ma rispettandole poi quando sono adottate. Questo è il senso di qualunque partecipazione collegiale a qualunque organismo che sia appunto collettivo: un'autolimitazione della propria sovranità. Ora, credo si faccia bene a

europea ed internazionale degli ultimi giorni ha consegnato probabilmente ai cittadini italiani un'Italia diversa da quella che eravamo abituati a vedere: un'Italia che conta

ritengo che la credibilità, che si conquista mantenendo fede agli impegni assunti in sede internazionale, giovi complessivamente al nostro Paese. Un'ultima considerazione riguarda il perché su questo provvedimento sia stata posta la fiducia. Sono pienamente d'accordo con le argomentazioni esposte in Aula ieri dal ministro Chiti. Per una legge elettorale, da altri voluta, al Senato vi è una situazione diversa da quella della Camera per cui quel che è stato fisiologico ed è fisiologico in tutti i Parlamenti, cioè una differenziazione tra alcune posizioni di minoranza, qui potrebbe diventare determinante per la vita dell'Esecutivo. A parità di consenso elettorale - ripeto - qui al Senato abbiamo una situazione che non ho difficoltà a definire patologica. Ed in presenza di tale difficoltà patologica, per una legge elettorale non da noi voluta, probabilmente l'unica mediazione intelligente, in grado di consentire ai senatori che volevano mantenere un distinguo o comunque delle differenziazioni rispetto al provvedimento proposto dal Governo era quella di

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea rifìnanzia la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, nonché la promozione di processi democratici in tali Paesi, anche attraverso la ricostruzione e riorganizzazione istituzionale e civile degli stessi, in linea con l'impegno assunto dall'Italia da più legislature e sotto la guida di Governi diversi. Le missioni rifinanziate dal provvedimento in esame sono ben ventiquattro, anche se l'attenzione si è focalizzata per lo più sull'Afghanistan e l'Iraq. Signor Presidente, oggi in quest'Aula il problema non è tra maggioranza ed opposizione, bensì all'interno della stessa maggioranza di centro-sinistra, che si trova profondamente divisa, spaccata da un tema tanto importante e delicato qual è la politica estera e di sicurezza. Una politica estera e di sicurezza, quella del Governo Berlusconi, portata avanti con coerenza per cinque anni e diretta soprattutto a contrastare il terrorismo, sia talibano sia iracheno, e porre fine ad un regime dagli effetti disastrosi, portando a termine il processo di pacificazione e di ricostruzione di quelle zone. Ritengo, anche a nome del Gruppo Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia, che la lotta al terrorismo rimane una priorità e non può consentire discontinuità; i nostri soldati si trovano in Afghanistan nel quadro di un impegno militare internazionale che prosegue oggi per portare pace, libertà, sviluppo e anche democrazia. Per quanto riguarda l'Iraq, l'attuale Governo non ha fatto altro che prendere atto di quanto aveva già deciso il Governo Berlusconi,

in coerenza con i princìpi che hanno guidato la politica estera del Governo di centro-destra nella sua lotta al terrorismo internazionale, ma non voterà la fiducia posta dal Governo sul provvedimento in esame innanzitutto perché non accettiamo il «papocchio impastato» dal centro-sinistra, che per l'approvazione di un provvedimento così significativo ed importante per la politica internazionale si avvale dello strumento della fiducia, l'utilizzo del quale dovrebbe essere di natura eccezionale. Inoltre, vorrei anch'io sottolineare, come è già stato fatto da tutti i colleghi che mi hanno preceduto, che l'utilizzo della questione di fiducia mortifica il ruolo centrale del Parlamento. Il Paese deve sapere che il nostro Gruppo è a favore della trasparenza. La nostra posizione su questo delicato e importante argomento, che la comunità internazionale saprà giudicare nel modo più giusto e appropriato, è univoca e favorevole al provvedimento in esame, così come manifestato anche dai colleghi della Camera dei deputati. Anche il mio Gruppo, quindi, in quest'Aula, condivide la posizione dei colleghi della Camera; tuttavia, non può concedere la fiducia ed il voto a questo Governo, che si è avvalso dello strumento della fiducia, direi quasi per estorcere, da 16 colleghi del centro-sinistra un voto che certamente in più occasioni hanno manifestato di non condividere. Ribadisco che noi siamo favorevoli, come più volte e in più sedi dichiarato, al finanziamento della missione in Afghanistan, ma non siamo favorevoli assolutamente a questo Governo per quanto riguarda tutto il suo operato ed in particolar modo quello sulla politica estera. Quello che vogliamo dire al Paese con forza è che siamo favorevoli al rifinanziamento delle missioni internazionali, ma al Governo non daremo mai, dico mai, il nostro voto di fiducia. Il Governo in questa occasione merita solo la nostra sfiducia per non aver accolto l'invito del centro-destra per un voto libero di tutti i senatori. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, oggi più di ieri la strada che dobbiamo percorrere, che il nostro Paese deve promuovere, è quella di una comunità internazionale che abbia fondamenta sullo sviluppo, la solidarietà tra i popoli e il rispetto del diritto internazionale, nonché dei principi dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione sul proprio territorio. A chiedercelo, ad imporcelo, è quell'articolo 11 della Costituzione che i Padri fondatori della nostra Repubblica vollero scrivere a dimostrazione della vocazione di pace del nostro popolo. Ed è tenendo presenti questi valori che l'Italia, di fronte alle gravi sfide che la comunità internazionale ha davanti, deve farsi promotrice della creazione di un ambiente di sicurezza globale, valorizzando i mezzi preventivi di risoluzione delle controversie. Tengo a sottolineare in tal senso che il Gruppo Per le Autonomie è fermamente e convintamente contrario all'uso della forza come strumento per la risoluzione dei conflitti internazionali. Anche per la lotta al terrorismo, una comunità di Stati di diritto possiede ben altri strumenti di risposta: la creazione di una polizia internazionale sotto la guida delle Nazioni Unite, i servizi segreti, interventi più mirati, la politica e la diplomazia. Lo affermo oggi come lo feci da questi banchi il 7 novembre 2001, quando, pur esprimendo profonda solidarietà nei confronti degli Stati Uniti per l'attentato alle Torri gemelle, ribadii il mio forte dissenso e il mio categorico no al ricorso alle armi per la risoluzione dei conflitti internazionali. La storia ci ha dato ragione: è cresciuto l'odio tra le culture ed è cresciuta la solidarietà fondamentalista nel mondo islamico. Per poter sradicare veramente e a lungo termine fenomeni che danno adito al terrorismo, infatti, si devono capire le ragioni che stanno nella contrapposizione tra il mondo ricco e sviluppato ed i Paesi poveri, destinati o all'immigrazione o alla rassegnazione, oppure al fanatismo e all'odio. Anche e soprattutto le religioni devono saper convivere pacificamente tra loro, senza rivolgere al loro interno l'attitudine inquisitoria e persecutoria. La cosiddetta guerra giusta o preventiva è e si è rivelata una strategia fallimentare e lo dimostra l'*escalation* di violenza che infiamma quotidianamente l'Iraq, l'Afghanistan e che in queste ultime settimane ha ridato fuoco alla polveriera del Medio Oriente. Oggi più di ieri è necessario il rafforzamento delle grandi organizzazioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite, ed un ruolo nuovo e rafforzato dell'Unione europea, perché solo un'Europa che parla a voce unisona può essere attore principale e determinante nello scacchiere delle crisi internazionali. È questa, assieme alla strada del multilateralismo, la vera ed efficace lotta contro il terrorismo e l'unico strumento per realizzare un equilibrato assetto multipolare, di equità e di giustizia sul piano internazionale. Onorevole signor Presidente, oggi in quest'Aula del Senato siamo chiamati a pronunciarci sul rifinanziamento delle missioni italiane all'estero; a titolo personale e da convinto cristiano mi permetto di ricordare che ho sempre votato contro il provvedimento che impegna le nostre truppe in scenari di guerra. Accolgo, e insieme a me tutti i membri del mio Gruppo, quindi, con favore la decisione presa dal Governo di ritirare il nostro contingente dall'Iraq, come peraltro previsto dal programma dell'Unione. La missione «Antica Babilonia», infatti, era nata in conseguenza di un intervento militare deciso in violazione delle norme di diritto internazionale. Pertanto, riconosciamo la diversità delle condizioni della presenza in Afghanistan, in coerenza con gli impegni multilaterali presi nell'ambito dell'ONU. Tuttavia, e lo dico con tutta apertura, ma anche come avvertimento per il futuro, ci auguriamo che quantomeno si realizzino le condizioni affinché il nostro Paese, d'intesa con il Governo sovrano di Kabul e con l'ONU, possa disporre il rientro delle nostre truppe anche dal territorio afgano. Positive sono in tal senso le verifiche, previste negli ordini del giorno, sulla missione internazionale e sugli obiettivi che il Governo italiano vuole portare avanti, assieme alla promozione di una nuova conferenza internazionale che favorisca il dialogo a livello regionale e sia volta alla ricostruzione economica e civile del Paese. Ritengo personalmente, e come Presidente del Gruppo Per le Autonomie, che questi aspetti rappresentino di fatto segnali di discontinuità della politica estera italiana rispetto al Governo Berlusconi. Accogliamo con favore che l'impegno militare dell'Italia in territorio afgano, nell'ambito della missione *Enduring* *Freedom*, sia stato limitato alla presenza di unità navali nel Golfo arabico. Tuttavia, richiediamo con fermezza al Governo Prodi la totale cancellazione della partecipazione italiana dalla succitata missione e che si impegni al suo superamento a livello internazionale, così come richiesto nell'ordine del giorno presentato da tutti i Capigruppo di maggioranza e da me stesso. La politica estera del Governo, a nostro avviso, deve prioritariamente valorizzare gli strumenti di prevenzione dei conflitti, di mediazione e di accompagnamento dei processi di pace.

Per concludere, onorevole Presidente, intendo preannunciare il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al Governo e, di conseguenza, al provvedimento. Il nostro, però, è un sì sofferto e per me, personalmente, è un sì condizionato all'appello di pace e di ripensamento sulla condizione afgana. È un sì che chiede il ritiro dalle azioni belliche e un sì fortemente condizionato dalla fiducia posta dal Governo. *(Applausi dai

Signor Ministro, onorevoli senatori, la fiducia al Governo Prodi, da parte nostra mai in discussione, accompagna però una vicenda molto difficile, quella delle missioni italiane all'estero, della nostra partecipazione in alcuni casi a vere e proprie guerre. Il nostro Gruppo che vede assieme Verdi e Comunisti Italiani ha manifestato con nettezza il proprio dissenso. Nel suo discorso d'insediamento, il presidente Prodi ha affermato senza tentennamenti che la guerra è sbagliata, che il terrorismo se ne alimenta e che le truppe dall'Iraq andavano ritirate. Un discorso che ha suscitato - mi creda, signor Ministro - molte speranze e molte aspettative, non solo in quest'Aula, ma soprattutto nel Paese, in quello straordinario movimento per la pace che è schierato con il nostro Governo. Allo stato attuale, però, parte di quelle speranze e di quelle aspettative sono deluse: voglio dirlo con chiarezza. Mi permetto di dire, per esempio, che il ritiro dall'Iraq sta avvenendo tardivamente, e soprattutto quasi in sordina, cosa incomprensibile. Come se dovessimo attenuare, in qualche modo, quella scelta giusta e coraggiosa, sicuramente il più dirompente atto di rottura rispetto a cinque anni di Governo delle destre. Il giorno dell'insediamento, il presidente Prodi ha detto una verità che tutti, tutto il mondo - anche quest'Aula - sa ma non dice: le guerre, appunto, alimentano il terrorismo. Infatti, dopo l'invasione dell'Iraq, il terrorismo si è allargato a dismisura, ha contagiato aree enormi del Medio Oriente, dove prima il terrorismo non c'era, fino a diventare, nella coscienza di tante donne e di tanti uomini di quei Paesi, uno strumento disperante e terribile, non so come definirlo, ma comunque uno strumento di identità. Quindi, una cosa spaventosa, più spaventosa dell'atto stesso, per alcuni versi.

Poco meno di un mese dopo l'attacco alle Torri Gemelle, il 7 ottobre 2001, gli USA hanno attaccato l'Afghanistan con la missione *Enduring Freedom*, una missione, checché se ne dica, feroce e illegittima, senza copertura ONU, che ha ucciso e uccide migliaia e migliaia di uomini, donne, bambini e anziani: civili ed incolpevoli. Signor Ministro, onorevoli senatori, se ne fossi capace vorrei veramente parlare non soltanto alla testa, ma al cuore di tutti noi. Fino a quando si continuerà a dare legittimità politica alla menzogna dell'aggressore aggredito, che pratica il terrorismo perché ha il diritto di difendersi dal terrorismo? Fino a quando si continuerà ad accettare l'esistenza di carceri, molte segrete, proprio sul territorio afgano - e non solo su quel territorio - in cui si pratica la tortura? Per quanto ancora non si dirà che il problema vero in Afghanistan è la povertà estrema, inenarrabile, indicibile, che il problema vero è un Governo fantoccio e corrotto, composto da personaggi che depredano il Paese, legato ai talibani, ai signori della guerra, ai trafficanti di oppio? Fino a quando si assisterà impassibili alla mattanza di afgani, di iracheni, di libanesi, usando la forza per imporre ciò che il diritto vieta? Si è incendiato tutto il Medio Oriente, si è messa in atto una guerra di religione e di civiltà, e l'Occidente ha rivendicato il ruolo di unica forza di diritto e di democrazia. Ma l'Occidente ha usato menzogne: ha detto che l'Iraq possedeva armi di distruzione di massa, ha detto che l'Afghanistan andava liberato dai talibani e alle donne andava restituita dignità, mentre nel frattempo apre un altro pericolosissimo fronte con l'Iran, ma nulla dice, ad esempio, è un esempio emblematico di quel che succede in Pakistan con il dittatore Musharraf. In nome di cosa l'Occidente si arroga il diritto di stabilire chi siano i buoni e chi i cattivi, quali dittatori fanno comodo e quali vanno eliminati? L'Occidente non ha diritti per stabilire la verità del mondo: della sua storia fa parte la spaventosa vicenda dell'Olocausto, nella sua storia c'è la bomba sganciata su Hiroshima, vicende che sono avvenute ad opera nostra, nella culla della civiltà e della democrazia, non in Oriente. L'Iraq non possedeva armi di distruzione di massa, il terrorismo non c'era, oggi c'è. In Afghanistan italibani sono più forti che mai, Al Qaeda non è stata sconfitta e il destino delle donne - e non solo delle donne, ovviamente - è stato rimesso nelle mani degli ulema, la polizia religiosa. La guerra in Afghanistan, signor Ministro, onorevoli senatori, è sbagliata. La nostra presenza lì non ha ragione di essere. Da qui il nostro dissenso, un dissenso politico, non di coscienza, non da anime belle! Un dissenso politico irriducibile. Eppure, nel frattempo, in politica estera - voglio dirlo, perché altrimenti la mia sarebbe solo una protesta inutile, sterile, arida - sono avvenuti fatti significativi di cui do atto al Governo e di cui sono contenta e orgogliosa, e assieme a me lo sono i compagni del mio Gruppo. alle prese di posizione del ministro D'Alema su Guantanamo e sul caso Calipari. A proposito, il senatore Castelli non dovrebbe strumentalizzare vicende tanto dolorose e l'Assemblea, tutta l'Assemblea, onorevoli senatori, dovrebbe impedirglielo. Quelle prese di posizione sono state il primo segnale di un recupero di autonomia nei confronti degli Stati Uniti. I primi commenti del presidente Prodi sulla questione israelo-libanese e il *summit* tenuto a Roma hanno rimesso in luce la vocazione

Nessun atto di prepotenza da parte del presidente Prodi, onorevoli senatori dell'opposizione: qui non c'era il rischio di non avere la maggioranza dei voti, ma che di voti ce ne fossero anche troppi, e che si utilizzasse il dissenso sulla guerra per inquinare la maggioranza che gli elettori hanno scelto e votato. Il sostegno delle destre non sarebbe avvenuto gratis, ci avrebbe diviso su una questione dirimente che è nel DNA, ne sono sicura, di tutto il centro-sinistra. Per questo, abbiamo esplicitamente avanzato al Governo la richiesta di porre la fiducia. Il Governo ce l'ha concessa e per questo lo ringraziamo: è il riconoscimento della legittimità delle diverse posizioni; è il sintomo della forza, non della debolezza dell'Unione. Sono, infatti, i deboli che prendono posizioni chiuse ed intransigenti; i forti sanno capire, ascoltare e accogliere le diversità. Il nostro voto di fiducia convinto è il segno della nostra piena appartenenza all'Unione. Ma, come il Governo sa, noi siamo gente testarda, continueremo a batterci per le nostre idee, vogliamo vedere i nostri tornare dall'Afghanistan. Non faremo sconti, ma saremo alleati leali su cui il Governo potrà contare. Insomma, per finire, dobbiamo operare per arrivare al tempo della pace, perché questo è il tempo della costruzione, della fine delle esclusioni, dei pregiudizi e delle divisioni; è il tempo della vita, che è cosa troppo preziosa per essere lasciata alle armi. Auguro, dunque, buon lavoro al Governo Prodi.

Signor Presidente, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori,

dalla cui lettura ho ricavato ragioni sufficienti per ribadire che il Gruppo dell'UDC conferma il proprio voto favorevole ideale al disegno di legge n. Ideale perché il Gruppo dell'UDC, come opposizione, è impedito a convergere con un voto aperto ed esplicito dalla procedura parlamentare che, stando a quello che abbiamo potuto ascoltare dalla senatrice Palermi, è stata imposta al Governo da alcuni *partner* della maggioranza. Si tratta di un vero e proprio capovolgimento di rapporto se il Governo riceve l'impulso e, vorrei dire, il *diktat* a chiedere il voto di fiducia per impedire convergenze dell'opposizione. Devo ripetere che il Gruppo dell'UDC, come ritengo gli altri Gruppi dello schieramento di opposizione, sulla politica estera, e quindi sulla politica della sicurezza che è implicita nella linea della politica estera, non porrebbe una pregiudiziale, una pregiudiziale, nei rapporti con il Governo, proprio perché siamo portatori della convinzione che sul terreno della politica estera debba essere sempre ricercata una linea di convergenza - come si usa dire - *bipartisan* o, forse, sarebbe preferibile dire, con una locuzione di qualche stagione politica passata, di unità nazionale. di unità nazionale. L'Italia è impegnata in alcune missioni estere; in questo ordine del giorno presentato dalla maggioranza se ne dà un giudizio positivo. Viene avanzata una riserva esclusivamente nei confronti dell'impegno assunto in Iraq e lo si discute sotto il profilo della legittimità e della legalità internazionale. Vorrei limitarmi a ricordare che l'Italia è intervenuta in Iraq soltanto dopo la prima risoluzione dell'ONU; quindi è vero che la decisione di intervento in Iraq è da attribuire a due Stati alleati (ai quali l'Italia, tuttavia, è legata per ragioni di politica internazionale che poi si riportano al grande capitolo della NATO),

Vorrei dire che, sia pure *a posteriori*, c'è stata una sanatoria di legittimità da parte dell'ONU, che è tornata ripetutamente a occuparsi e a definire una propria posizione, anche unanime, con successive risoluzioni, dalla 1500 del 14 agosto 2003 fino alla 1546. Vorrei far presente - nessuno credo possa disconoscere questo dato - che la realtà politica e anche istituzionale dell'Iraq oggi è ben diversa da quella rappresentata e raffigurata dal regime di Saddam Hussein. C'è un Governo di unità nazionale, un Governo di coalizione, c'è un primo tentativo di far stare insieme, in un'area difficile e complessa (ma tutta la storia dell'area mediorientale, dalla caduta dell'Impero ottomano è storia di travagli, che ha coinvolto, a volte anche tragicamente, il mondo occidentale e l'Europa),

elemento fondamentalmente positivo per la costruzione dell'equilibrio in tutta la regione. Questo modello dovrebbe essere esemplare per tutta l'area: una convivenza, anche in termini federalistici di tre etnie, di due religioni, di due culti all'interno della medesima religione, che tradizionalmente si sono sempre avversati. sempre avversati. La pace politica in Iraq è la premessa per tentare di costruire la pace in tutta quell'area, che vediamo oggi sottoposta a convulsioni drammatiche. Ma ritorno all'ordine del giorno della maggioranza.

per costruire la pace, fedelmente e coerentemente al nostro impegno costituzionale rappresentato nell'articolo 11. Ma questa è una linea di fondo e di continuità - l'ho detto ieri e lo ripeto - della politica estera italiana da De Gasperi fino ai nostri giorni; al di là della diversità di formula e carattere politico, da De Gasperi a Berlusconi, attraverso tutti i Presidenti del Consiglio e i Ministri degli affari esteri che si sono succeduti dal 1946 fino al 2006. È una costante, anzi, della politica estera italiana nel quadro della solidarietà con gli alleati, dei quali fondamentali sono gli europei. È un'invocazione a costruire l'Unione Europea; è stata un'intuizione di De Gasperi, a cui si è lavorato in questi cinquant'anni, un'intuizione ancora non consacrata né in realtà istituzionale, né in realtà politica.

Omaggio ai nostri amici alleati francesi, ad una Nazione la cui storia e cultura compenetrano profondamente la storia e la cultura italiana, ma da De Gaulle in poi da De Gaulle in poi abbiamo sempre dovuto misurare uno scarto, una differenza fra la politica estera francese, fra la concezione che hanno i francesi dell'Unione, dell'unità europea, e quella portata avanti dall'Italia in ogni tempo. Non sono elementi che intendo evidenziare per stabilire un limite rispetto al quale tornare indietro, ma un limite rispetto al quale andare avanti. L'unità europea non è ancora una realtà: dobbiamo costruirla. Certo, se fosse se fosse stata realizzata l'intuizione di De Gasperi avremmo oggi un esercito europeo, allora gli interventi dell'Italia e dell'Europa unita per ottenere sempre una politica di sicurezza, non soltanto in Europa, ma nel quadro mondiale, laddove si giocano interessi vitali dell'umanità, prim'ancora che della nostra Nazione, sarebbero pacifici.

perché il voto che avremmo voluto esprimere sul disegno di legge n. 845 (come è stato dato alla Camera, e le motivazioni sono state, per quello che ci riguarda, felicemente espresse dal presidente Casini, e quindi mi limito a riproporle) riflette ragioni di convergenza su una politica che noi consideriamo debba rappresentare il tema del bene comune. Possiamo dividerci, distinguerci su tutte le altre questioni, possiamo anche discutere e dibattere il modo di impostare la politica estera, ma non possiamo non avere il senso di una tendenziale unità nazionale su questo terreno. Ecco perché riconfermo che noi votiamo contro la fiducia al Governo Prodi nella forma che abbiamo già realizzato nel voto di ieri sera, il cui esito, peraltro, spiacevolmente è stato controverso. *(Applausi dai

Ad ascoltare gli interventi dei colleghi della sinistra è difficile, signor Presidente, rimanere indifferenti;

stata la contrarietà alle missioni di qualsiasi tipo che utilizzassero personale militare. La conclusione unanime è stata, viceversa, il voto alla fiducia su un provvedimento che rifinanzia

Per comprendere tale meccanismo, dobbiamo risalire ad Antonio che nemmeno nell'orazione a Cesare fu tanto abile da partire con una premessa e finire con l'esatto opposto. andiamo a vedere i termini con cui si è ragionato; è probabile che siano stati sfogliati bene sia lo Zingarelli sia il Devoto-Oli, perché sono stati utilizzati tutti i sinonimi e tutti i contrari.

riferito al rifinanziamento delle missioni militari. Guardate bene: c'è un prefisso nel termine "rifinanziamento". Dove sta la discontinuità? È difficile far quadrare il cerchio.

confessare. Il Governo pone la fiducia. Ministro Parisi, la fiducia è uno strumento che ha un senso, una logica e una funzione. Se mi passa il termine, la fiducia è un po' una purga, una purgazione. Il Governo deve accantonare degli emendamenti, delle manovre ostruzionistiche, ha necessità di chiudere quel provvedimento, *ergo* pone la fiducia. Ma non si può chiedere la fiducia, o meglio utilizzare una purga, per combattere il mal di pancia, perché qui si tratta di mal di pancia interno alla compagine che governa. Il mal di pancia si poteva preventivare, ministro Parisi, nel senso che lei ha una maggioranza mai composta, per essere composti nel modo di esporre. Il DNA dei comunisti canonici esiste ancora in gran parte di questa maggioranza, che considera lo Stato come una sovrastruttura da abbattere per raggiungere l'utopia. Loro hanno sempre combattuto tutti gli organismi che rappresentano lo Stato. I bersagli di quella cultura sono sempre stati gli organismi dello Stato; sono stati la magistratura, la polizia, le stesse istituzioni. Figuriamoci poi i militari! Come può vedere questa cultura di sinistra il sistema militare? La mano armata dello Stato.

dove gli Stati sono governati da tagliatori di teste. Nemmeno questo, per la loro cultura, giustifica l'intervento di una comunità sovranazionale, in ogni caso, che intende tendere una mano a quei popoli, ai cittadini soggiogati in quei Paesi. Ma l'apoteosi in quest'Aula vi è stata con un comportamento di somma ipocrisia. Quando qualche oratore ha ricordato gli eroici militari caduti per difendere e garantire il nostro Paese,

al grido e alle scritte di «dieci, cento, mille Nassiriya»! Ma qual è il loro riferimento? È il rispetto delle istituzioni, dei nostri organismi, della nostra struttura di difesa o è quella parte

Per governare il Paese servono probabilmente altre formule, e non saranno le fiducie ripetute che lo terranno assieme e faranno da cemento.

Questo pensiero di Ghandi mi pare squaderni nel dibattito politico un tratto fondamentale della nostra identità. Democrazia e diritti umani non vivono nella imposizione e nella coercizione di missioni di guerra unilateralmente imposte da un comando imperiale, tanto più devastante quanto più è in crisi di modello e di egemonia. Essi vivono nelle missioni di pace, che alludono a cooperazione, a diplomazia preventiva, a dialogo, a solidarietà. Il pacifismo non vive di torsioni politiciste né di gabbie istituzionali, come ci insegna ogni giorno da molti anni la senatrice La pace non è solo assenza di guerra: è un pieno di opere, di impegno, di passione. È un saper fare quotidiano, un coagulo di soggettività plurali, di percorsi verso un mondo non violento fatto di mille rivoli carsici: dalle obiezioni di coscienza e fiscali alla riduzione delle spese militari, alle riconversioni dell'industria bellica, dal commercio equo e solidale alle cooperazioni internazionaliste tra popolo e popolo. Ci ammoniva padre Balducci dall'Abbazia fiesolana: "Non c'è pace senza giustizia". essere in definitiva ripensata la stessa collocazione geopolitica del nostro Paese. Deve essere rielaborato il sistema complessivo di intervento, rifondando una politica estera che sfugga al nodo scorsoio della guerra preventiva globale. La vera posta in gioco quindi è una nuova politica estera, che parta dal dramma israelo-palestinese, un dramma che incide a sangue le nostre carni di Paese euro-mediterraneo. Il nostro giudizio è che questo Governo ha segnato, in poche settimane, passi importanti di un cambiamento di strategia. Il ruolo ancillare del Governo Berlusconi verso la guerra preventiva globale di Bush è già un incubo che si va dissolvendo. L'Europa ridiventa centrale. Roma è stata sede della Conferenza internazionale. Da qui può riprendere il cammino di pace che può condurre alla sicurezza dello Stato di Israele ed alla costruzione dello Stato palestinese. Uno Stato non in forma di *Bantustan*, di poveri ghetti blindati dall'esercito di occupazione, ma uno Stato fondato su terre continue, continue, contigue e autonome e con una capitale comune, Gerusalemme, che torni ad essere la città meticcia della condivisione culturale, dove le differenze arricchiscono i rapporti tra popoli diversi ma uguali. Questo Governo tenta di ridare un ruolo alle Nazioni Unite, una struttura indispensabile per il governo diplomatico dei conflitti, che è stata annichilita, mortificata, cancellata dal Dipartimento di Stato americano con l'attiva complicità del Governo Berlusconi. Anche il riconoscimento del diritto di cittadinanza ai migranti basato sulla residenza; le leggi sull'asilo e sul diritto di voto in avanzata preparazione; il riconoscimento del diritto a essere con noi, uguali a noi, a 350.000 immigrati che il lavoro nero e sommerso rendevano clandestini, sono splendidi atti di politica internazionale e, insieme, interna perché parlano di noi, di come immaginiamo la nostra società, noi stessi, le nostre città future, il nostro Stato di diritto. Blindati ed emergenzialisti, come per cinque anni ci hanno voluto le destre xenofobe, o capaci di essere transnazionali, cittadini del mondo, fieri della nostra civiltà giuridica? Né è lecito sottovalutare la decisione, tutt'altro che facile o incontrastata, di far rientrare tutti i militari italiani dall'Iraq. Il rientro totale delle truppe italiane è un passaggio importante, di inversione di tendenza, sia per quanto concerne gli equilibri geopolitici (la costruzione di un multipolarismo dinamico), sia per quanto concerne l'impegno pacifista, che ha visto coronati tre anni di mobilitazione continua, fondata proprio su una visione globale e plurale. Sì, due aggettivi, globale e plurale; perché il pacifismo contemporaneo o ha questa identità o non è, e non riesce più a costruire percorsi e politiche di pace. Il risultato attuale sulla missione militare e di guerra - ripeto, di guerra - in Afghanistan è certamente molto meno nitido. Rifondazione Comunista-Sinistra Europea ribadisce il suo giudizio negativo su questa missione. Da qui è nata anche, certo, la sofferta divisione al nostro interno,

Abbiamo voluto invece, con un dibattito serrato e non banale, contestare quello che a me è parso un errore politico grave, che ha inciso anche sulla compattezza della nostra comunità, che è interamente pacifista. In un passaggio per noi aspro, difficile, abbiamo sottoscritto sull'Afghanistan quello che ho chiamato «un compromesso dinamico». Lo chiamo compromesso, perché noi sappiamo dire la verità: non chiamiamo vittorie quelle che vittorie non sono. "dinamico", perché per tutti noi e per il movimento pacifista l'obiettivo strategico rimane, senza ripensamenti, quello di un disimpegno totale dalle operazioni militari e di una riconversione totale della missione in direzione cooperativa e diplomatica. Certo, l'esito è anche nelle mani dei movimenti di massa. Non crediamo che esistano governi "amici", a cui i movimenti e i conflitti debbano essere subalterni, né pensiamo che i movimenti possano essere, dai dirigenti politici, imbavagliati o subordinati alle tattiche di governo. I movimenti non sono l'abito buono del dì di festa, che vanno rinchiusi nell'armadio quando la politica si fa seria e di Palazzo, perché sono essi movimenti la leva della ricostruzione dialettica di uno spazio pubblico che sappia fuoriuscire dalla crisi della politica contemporanea. La sfida che abbiamo posto a noi stessi è di mantenere salda la barra di navigazione, di dimostrare, nei fatti, la possibilità concreta di operare, anche dall'interno del Governo e della maggioranza, come forza che è parte dei movimenti e insieme capace di aprire dei varchi che consentano ai movimenti di avere efficacia, conquistando obiettivi politici ogni giorno. Non possiamo semplificare questa complessa dialettica sull'altare di vessilli identitari o puramente testimoniali. il nostro sì oggi è frutto di un giudizio. Un giudizio buono, molto buono su questo Governo. Il Governo dell'Unione non è per noi una camicia di forza, ma un'occasione, uno straordinario passaggio per l'alternativa. In maniera criticamente unitaria, ci facciamo garanti del suo profilo riformatore, cioè in definitiva - avremmo detto con vecchio linguaggio - delle aspettative e delle speranze delle masse popolari. Siamo convinti che il clima di rinnovata attesa e di rafforzamento dello spirito civico, che cresce nel Paese, siano lievito di questa maggioranza. Chi ne attende il disfacimento, sarà un impotente profeta di sventure. Termino con le parole di Pietro Ingrao: «Se nel tragico scenario dell'incendio mediorientale non ci si adopera per costruire una solida iniziativa del Governo, sostenuta da un'Unione compatta, mancheremmo sulla prima questione cruciale che ci troviamo di fronte dopo la vittoria elettorale, rischiando, addirittura, di dare carte allo sconfitto Berlusconi». Senatrici e senatori, Rifondazione Comunista sa bene che non ce lo possiamo permettere; questo è il nostro azzardo, questa è la nostra sfida, ma - riteniamo - questo è per l'appunto il sale della politica, della politica vera.

abbiamo ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi che si sono succeduti nel corso di questo dibattito, per giungere alla conclusione che è difficile comprendere quale sia la linea

dove si rileggono molti dei passaggi che in Parlamento si sono ascoltati. Si capisce che il senso della discontinuità - che è diventato lo *slogan* di questo dibattito si ritrova in molte delle affermazioni che in quell'ordine del giorno richiamano il multilateralismo come punto di riferimento di tutta la linea politica italiana. infatti, arriva ad un delirio di multilateralismo che francamente abbiamo trovato poche altre volte, impegnando il Governo ad operare in sede ONU per formare forze militari dell'ONU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 Su questo delirio di multilateralismo, che rappresenta la sola discontinuità verso la politica estera e che nulla ha a che vedere con un rifinanziamento delle operazioni militari, vorrei la vostra attenzione: il multilateralismo è sostanzialmente l'organizzazione delle Nazioni Unite. Spesso, molto spesso, il multilateralismo è stato usato nel dibattito di politica estera come la foglia di fico dell'impotenza delle forze internazionali o delle forze politiche che all'ONU ricorrono nella misura in cui affidano ad altri, ad un ente virtuale,

si è ben guardato dal parlare di multilateralismo. Il Ministro ha parlato di un'operazione di una coalizione di volenterosi in cui auspica di vedere molte Nazioni europee, certamente non sotto l'insegna dell'ONU, nella speranza di giungere ad una risoluzione, senza l'appoggio NATO che è certamente un'altra organizzazione multilaterale. Quando nella pratica, nella realtà, nella concretezza della politica estera si arriva a fare una scelta, si riconosce che le coalizioni multinazionali sono quelle maggiormente in grado di incidere nelle vicende della politica internazionale. al di là di questa ricerca di discontinuità, vi è la fiducia che è stata richiesta al Senato. Una fiducia sulla quale il ministro Chiti ci ha dato un'ampia spiegazione - a dire il vero, nemmeno chiesta da noi - che evidentemente era rivolta all'interno della maggioranza. Devo dire che quanto più l'onorevole Chiti parlava, quanto più il dibattito proseguiva in quest'Aula, tanto meno ho compreso le ragioni di questa fiducia.

dei pacifisti, sebbene il senatore Russo Spena giustamente dichiari che pacifista è tutto il centro-sinistra. La realtà è che da oggi vi è un nuovo soggetto politico all'interno di quest'Aula che ha avuto, attraverso la fiducia, la legittimazione ad operare, ad agire, a proporre. Lo si è visto all'inizio del dibattito di ieri, quando sono intervenuti più o meno tutti i rappresentanti di questo nuovo soggetto politico, in una posizione isolata; soli, non certo davanti ad un uditorio attento da parte del centro‑sinistra. Nell'onestà intellettuale che va loro riconosciuta, non hanno fatto sconti al Governo

che ritroveremo probabilmente all'inizio del 2007 quando si discuterà il rifinanziamento delle missioni militari all'estero. Hanno decisamente dichiarato

non è che non abbiano ottenuto nulla. Il senatore Martone, in una sua dichiarazione, ha ricordato un altro passaggio di quell'ordine del giorno (trascurato nel dibattito e nemmeno difeso da chi lo ha lo ha presentato) in cui si impegna il Governo alla costituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio permanente delle missioni internazionali di pace che consentirà al Parlamento, attraverso missioni *in loco* e avvalendosi del contributo di personalità della società civile e di operatori umanitari impegnati nelle aree interessate (faccio una scommessa, ma credo che il primo nome sarà quello di Gino Strada), di verificare in maniera costante e puntuale il perseguimento degli obiettivi definiti dal Parlamento. In

consulenza di personalità della società civile e di operatori umanitari impegnati nelle aree interessate. Si tratta di un nuovo modo di procedere nella politica estera, forse anche questo multilaterale, che però ci preoccupa perché vuol dire che il nuovo soggetto politico che si è formato all'interno del centro-sinistra e che è anche un soggetto politico - visti i numeri che si muovono in quest'Aula - diventa determinante per ogni azione di politica estera che questo Governo andrà a l'arma puntata contro il Governo perché alcune posizioni pacifiste radicali vengano, in qualche modo, riconosciute o addirittura possano influire sulle decisioni del Governo. Ed è di una posizione talmente radicale che si è manifestata ancor di più durante l'audizione del rappresentante speciale di Kofi Annan in Afghanistan, perché questo messaggio dell'ONU, questo credere nel multilaterale va bene a condizione che

ormai al di fuori di un dibattito che vive di realismo e di pragmatismo. La nostra preoccupazione, nel verificare che attraverso il voto di fiducia avete costituito questo nuovo gruppo politico, è che gli interessi nazionali, da questa

dei nemici di Israele e delle voci di Hamas e di *hezbollah*, quando andremo a discutere della forza di interposizione in Libano, augurandoci che si arrivi presto ad un cessate il fuoco. Una forza di interposizione che - ricordiamo - non deve andare né a Gaza né in Cisgiordania perché ha una funzione unica, che è quella di aiutare il Governo libanese a disarmare i terroristi di *hezbollah*. Con la fiducia il Governo ricrea una nuova e diversa posizione. E allora noi, che avevamo votato, fino all'articolo 1, anche in Commissione, con la convinzione profonda di chi appartiene a questo schieramento politico, quello di un mondo che crede nella libertà e nell'impegno del proprio Paese all'estero, che ha una forte cultura e un senso dello Stato e delle istituzioni, abbiamo votato a favore, senza nessun patteggiamento, al limite senza che ci venisse chiesto. Ne terremo nota. Continueremo in questo nostro comportamento, che appartiene al nostro DNA ed alla nostra cultura. Lasciamo al Governo la responsabilità di aver ceduto al ricatto di di aver ceduto al ricatto di questo gruppo minoritario all'interno del centro-sinistra. La nostra posizione è chiarissima: la fiducia ad un Governo Prodi, che rinuncia agli interessi nazionali nelle azioni di politica estera, non potrà mai vedere il nostro voto favorevole.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, come hanno ben spiegato i colleghi che da questi banchi sono intervenuti nella discussione, l'atteggiamento negativo di Forza Italia dipende essenzialmente dal fatto che, ponendo la questione di fiducia, il Governo ci impedisce di ribadire anche col voto la nostra piena e convinta adesione al rifinanziamento delle missioni internazionali di pace delle nostre Forze armate. Se c'è logica nei fatti politici, se c'è rapporto tra effetto e causa, questa è una vittoria politica della sinistra radicale. Altro che sinistra folcloristica, se riesce, come concretamente riesce, ad impedire alla metà del Senato di sostenere col voto l'opera meritoria e rischiosa dei nostri militari. Ma la vittoria dell'estrema sinistra è anche - prendetene atto, onorevoli colleghi - una sconfitta del resto della maggioranza, perché il ricorso alla fiducia come unico mezzo per evitare il tracollo della coalizione e, più ancora, il convulso dibattito interno che lo ha determinato ci hanno dato la prova provata - colleghi del centro-sinistra - che voi non avete una politica estera condivisa. E non l'avrete neppure dopo il voto, perché rimarrà comunque il dissenso motivato e decisivo di alcuni senatori, come rimarrà il dissenso, che ci è ben noto, di importanti settori del vostro elettorato, a meno che non si siano sciolte come neve al sole le folle pacifiste che invasero le piazze d'Italia anche contro la missione NATO a Kabul. Voi, dunque, non avete una politica estera condivisa. E poiché, come diceva Don Sturzo, senatore Colombo, la politica estera è la politica, voi non avete una politica. Cosicché siete costretti a muovervi come il cavaliere inesistente: una vuota armatura di potere dentro la quale, di volta in volta, problema per problema, risuona solitaria una voce, sia pure quella seria e impacciata, che abbiamo sentito ieri, del ministro Chiti. Martedì avete imposto la fiducia sugli inasprimenti fiscali e le cosiddette liberalizzazioni; oggi la imponete su cose terribilmente più serie: più serie: non vi sembra di cogliere tra l'una e l'altra un vuoto di iniziativa politica che prima o poi finirà per ingoiarvi? Conosciamo bene le vostre divisioni interne e tuttavia non riusciamo a spiegarci la passività con cui le subite, fino al punto da lasciar cadere nel nulla anche le più alte e insospettabili esortazioni al dialogo. Nei giorni scorsi abbiamo sentito esaltare, anche da scranni elevati - non il suo, presidente Marini - le virtù democratiche dell'autosufficienza; vi ricordo che, in un Paese diviso a metà dalle elezioni, voi vi siete già presa la responsabilità di scegliere unilateralmente i Presidenti di Senato e Camera, precludendoci di fatto la possibilità di una successiva convergenza sul nome del nuovo Presidente della Repubblica. Così, in base ad una autosufficienza che trascura perfino le funzioni di garanzia e rappresentanza generale di quei vertici istituzionali, voi avete prodotto una grave lacerazione politica e istituzionale, che nuoce alla vitalità democratica dell'intero Paese. Paese. Non solo, ma ora, procedendo a colpi di fiducia, voi estendete questa lacerazione alla dialettica parlamentare, insidiando gli stessi poteri d'indirizzo e controllo del Senato della Repubblica. Lasciatemi dire, col massimo rispetto, onorevoli colleghi della maggioranza, che in questa condotta io non riesco a vedere neppure l'ombra della grande tradizione parlamentare della sinistra italiana e dei cattolici democratici italiani. Avanti ieri si è tenuto a Roma un importante vertice internazionale che noi giudichiamo positivamente e che comunque ha registrato l'impegno fattivo del nostro Governo per rompere il ciclo della violenza e ricondurre il Medio Oriente sul sentiero della pace. Vi chiedo soltanto: cosa dovrebbe pensare un osservatore internazionale che, dopo avere apprezzato quell'impegno, vede ora lo stesso Governo impedire il voto favorevole di mezzo Senato a missioni di pace già in pieno svolgimento? La risposta è scontata: un Governo così non è credibile e toglie affidabilità al nostro Paese. Per questo contestiamo la richiesta di fiducia, ma allo stesso tempo condividiamo totalmente il rifinanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali per il mantenimento o il ripristino della pace. Ciò perché esse sono in perfetta continuità con gli atti di Governo che abbiamo deliberato negli ultimi cinque anni e sono in sintonia con le nostre scelte di fondo per l'Occidente, per l'unità europea, per l'Alleanza atlantica, per la storica amicizia con gli Stati Uniti d'America. Ma la stessa convinzione con cui sosteniamo la missione in Afghanistan ci obbliga ora, ministro Parisi, a considerare scrupolosamente, e col proposito di prevenirli, i gravi e crescenti rischi cui solo esposti i nostri militari. Mi limito, per brevità, a ricordare che in un Paese ancora fragile sul piano politico, della sicurezza e dell'ordine pubblico

si stanno moltiplicando gli attentati di ogni genere. In particolare, quelli con uomini bomba sono passati, dai 7 del periodo 2002-2004, ai 21 del 2005, ai 33 del primo semestre di quest'anno. Contemporaneamente, si infittiscono i messaggi più temibili contro gli europei, come quello di Al Zawahiri del 22 giugno, quello dei talibani del 16 luglio e quello di ieri dello stesso Al Zawahiri, che chiama espressamente la *Jihad* a combattere l'aggressione in Afghanistan. Bastano questi dati, signor Ministro, per farci dire che il nostro contingente in Afghanistan è esposto ad una minaccia terroristica potenzialmente più intensa, più mirata e distruttiva di quella che ha dovuto fronteggiare, a durissimo prezzo, l'altro contingente in Iraq. Perciò, vi chiediamo con forza di ampliare in ogni possibile modo i margini di sicurezza e la capacità operativa dei nostri militari, sia attraverso le dotazioni tecniche, sia attraverso le regole di ingaggio. Tra l'altro, e concludo, Presidente, sarebbe un modo né retorico, né banale per onorare la memoria di tutti i nostri caduti in missioni di pace. Su questo vi assicuriamo il nostro incondizionato

anche se oggi rifiutate la massima copertura parlamentare alla nostra missione, piegandovi alle ragioni più dannose delle scontro politico e a mediocri interessi di parte.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, mi sono chiesta più volte, nel corso di queste ultime concitate giornate di lavoro, riflettendo sulle questioni di merito e sulle questioni politiche che abbiamo affrontato, se noi tutti - maggioranza, opposizione e Governo - non abbiamo agito troppo stretti sulla contingenza. Lo voglio dire adesso nell'esprimere piena e convinta fiducia al Governo su questo provvedimento che la quasi totalità dell'Unione condivide e - vorrei aggiungere - anche la quasi totalità del Senato, visto l'esito unanime del voto in Commissione. Ciò, a parere dell'opposizione, rende paradossale e figlia di una concezione autoritaria del Governo l'apposizione del voto di fiducia (sorvolo sugli striscioni);

si afferma che il Governo non è legittimato, perché se non avesse posto la fiducia, avrebbe denunciato di non essere autosufficiente su una questione di politica estera e avrebbe denunciato cioè la propria fine. Vi sono, in tal senso, molte dichiarazioni di autorevolissimi esponenti dell'opposizione. Sta in questa contraddizione, senatore Mannino, in questa contraddizione e non nel discorso del ministro Chiti, il labirinto. Però, se io denuncio la contraddizione e voi evocate il labirinto, forse il motivo sta nel fatto che stiamo ragionando guardando troppo da presso e solo a ciò che sta qui ed ora sotto i nostri occhi. nostri occhi. Credo per davvero che nella situazione data solo l'apposizione del voto di fiducia permette di dare espressione del dissenso dei singoli - dei singoli, senatore Pisanu, non di un'intera forza politica - e di rappresentarla come è, legittima, di ospitarla nella coalizione e, insieme, di controbattere alla vostra argomentazione che tutto questo mette in discussione la solidarietà della maggioranza e la fedeltà al Governo. È un paradosso?

nuovo per il nostro sistema istituzionale e politico, di come stanno al mondo delle istituzioni, in un sistema bipolare, coalizioni che inevitabilmente hanno dentro di sé sensibilità diverse, soprattutto su temi sensibili quali la pace, la guerra, la vita È stato già così, senatore Pisanu, con il Governo Berlusconi, su una questione centrale di politica estera, come il voto sulla Costituzione europea, che segnò il dissenso non di singoli, ma di un'intera e importante forza politica che componeva la coalizione di centro-destra! E non ci furono dissensi, senatore Pisanu, autorevolissimi, anche di Ministri, sulla legge n. 40 del 2004 o sulla riforma elettorale? E forse questo condannò quel Governo e ne decretò la fine? Non uso questi esempi per spirito polemico, non mi importa: voglio capire, e voglio capire insieme, senatore Pisanu. Pisanu. Secondo me, il punto è che ancora non abbiamo trovato - non ci siamo neanche sforzati di trovare - la cifra nuova con cui ordinare i rapporti tra coalizioni e nelle coalizioni in un sistema bipolare. E anche questo fa gravare fa gravare su di noi la responsabilità del fatto che la lunga transizione politica italiana non si è conclusa. Il vostro reclamare di poter votare è pienamente legittimo, ma obbliga, non è gratis. Obbliga a considerare che, se ci sono questioni essenziali per il Paese, sulle quali l'opposizione voglia concorrere alla decisione comune, ciò obbliga e costringe a prescindere dalla polemica strumentale e dalla demagogia. Non lo dico, ovviamente, solo in senso a noi favorevole, senatore Guzzanti. Sono sincera: l'abbiamo conosciuta quella tentazione durante gli anni del Governo Berlusconi e alcune volte vi abbiamo ceduto. I colleghi che mi hanno preceduto, in tanti, hanno espresso in discussione generale le ragioni del nostro consenso a questo provvedimento, mettendo in evidenza la discontinuità che esso produce nelle scelte di politica estera del nostro Paese, e hanno fatto molto bene. Non voglio ripetere quegli argomenti, ma li voglio avvalorare, attribuendo a ciò che in questi giorni è avvenuto a due passi da qui, e cioè alla Conferenza di Roma, esattamente il peso e il significato di una riconoscibile, e ormai direi riconosciuta, in sede internazionale, politica estera italiana protagonista e non più subalterna, segnata dalla ricerca di soluzioni pacifiche al conflitto mediorientale. Infatti, non si tratta tanto del ritiro dall'Iraq, sul quale, sia pure senza affannarsi e con qualche ipocrisia, il Governo Berlusconi conveniva: la novità e la discontinuità stanno assai di più nella ritrovata autonomia, nel riferimento all'Europa, pur nella confermata saldezza delle relazioni con gli Stati Uniti e della collocazione NATO. Da questo derivano il ritiro dall'Iraq e la Conferenza di Roma. E non è un caso, per me, che di tutto ciò in quest'Aula, in questa discussione, non vi sia stato quasi traccia, tranne che nell'intervento del senatore Pisanu. Lo dico ai colleghi dell'opposizione, ma lo dico con la stessa forza ai nostri dissidenti dell'Unione: è come se l'osservatorio del Senato ancora una volta, come ho detto all'inizio, consistesse di un obiettivo troppo piccolo rispetto alle grandi questioni nazionali e internazionali. Ora non so se il senatore Guzzanti abbia trovato carino quello che ho detto; a me pare una faccenda tremendamente seria, come diceva Majakovskij, che richiede un gran lavoro, piuttosto che grandi strepiti. È la fatica e - come dice la senatrice Soliani - anche la grande bellezza della politica. Il Gruppo dell'Ulivo, colleghi, voterà sì, convintamente.

dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. Vorrei comunicare all'Aula che

il presidente Matteoli. Mi permetto, Presidente, di far presente un refuso, che sicuramente ci sarà, e che incide sull'onorabilità del presidente Marini, che sappiamo tanto corretto ed imparziale.

Ildisegno di legge in esame si compone di un unico articolo che prevede l'abrogazione di due decreti-legge in tema di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas, in quanto su tali provvedimenti, che pure rispondevano a problematiche reali, si è espressa negativamente la Corte di giustizia europea. Auspico pertanto l'approvazione del disegno di legge in esame da parte di questa Assemblea e chiedo alla Presidenza

siamo alla vigilia del decreto Bersani sull'energia ed è dunque importante riflettere sul passato per capire come potremmo meglio muoverci in futuro. L'inizio del processo di privatizzazione dell'energia elettrica e del gas naturale in Italia si può far risalirealla direttiva europea 96/92/CE del dicembre 1996, concernente le nuove norme per il mercato interno dell'energia elettrica. Con tale direttiva si stabiliscono le regole per la liberalizzazione dell'energia elettrica sul mercato europeo nella prospettiva di conseguire un mercato concorrenziale e non discriminatorio per quanto riguarda obblighi e diritti delle imprese elettriche. In sostanza, si prefigura un sistema di reti nazionali di trasmissione dell'energia interconnesse tra loro, sulle quali deve essere garantito il libero accesso ai produttori e ai fornitori di energia elettrica, in modo da permettere loro il raggiungimento degli utenti finali.

Poiché il processo di liberalizzazione ha avuto in Italia un impulso più forte che in altri Paesi europei, si è prodotta un'asimmetria con quei Paesi che hanno saputo proteggere in maniera più efficace le proprie imprese ed è rimasta irrisolta la questione, estremamente rilevante, la questione, estremamente rilevante, dell'ingresso massiccio di società europee nel nostro mercato nazionale per acquisirvi società. Il fatto puntualmente si è verificato nel maggio 2001,

del capitale sociale di imprese operanti nei settori dell'energia e del gas quando tali partecipazioni siano acquisite da imprese pubbliche non quotate in mercati finanziari regolamentati e che beneficiano nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante. Con la sentenza del 2 giugno 2005 la Corte di giustizia europea ha dichiarato che, mantenendo in vigore il decreto-legge n. 192 del 2001, convertito dalla legge 301

infatti, il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, con il quale si circoscrivevano i limiti all'esercizio del diritto di voto nelle deliberazioni assembleari alle imprese pubbliche titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, a condizione che lo Stato interessato abbia avviato le procedure di privatizzazione di tali imprese e abbia concluso accordi con lo Stato italiano volti a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato La Commissione europea ha ritenuto che, anche così emendata, la legge italiana non fosse conforme alla sentenza della Corte. Inoltre, la Commissione ha specificato che i requisiti di reciprocità reciprocità si riferiscono esclusivamente alla fornitura del servizio interessato e non riguardano la proprietà d'impresa o l'esercizio dei diritti derivanti da tale proprietà. Quindi, a difesa delle imprese italiane rimane al momento solo il comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, relativa al riordino del settore energetico, il quale prevede che: «Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione Europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati». In conclusione, al punto in cui siamo giunti in questa complicata vicenda vicenda i comportamenti dei vari Paesi europei sono orientati in senso protezionista e mettono in campo un'efficace tutela dei settori strategici nazionali, mentre in Italia ciò non è avvenuto e le imprese italiane risultano così esposte alle incursioni di società straniere ed al rischio della subalternità di fronte all'affermarsi di oligopoli stranieri. Si impone, quindi, un ripensamento delle politiche di liberalizzazione dei settori energetici, sia in rapporto al contesto internazionale che in rapporto al ruolo che questo Paese pensava di poter svolgere nel mercato internazionale e, infine, in rapporto alle politiche complessive di sviluppo industriale del nostro Paese. Riteniamo pertanto urgente la difesa dell'interesse nazionale e che venga fatto valere il principio di reciprocità, poiché quello dell'energia è un settore di rilevanza strategica nazionale sia rispetto strategica nazionale sia rispetto alla capacità produttiva e concorrenziale delle imprese, in particolare quelle manifatturiere, sia rispetto ai cittadini, sui quali si scaricano costi superiori a quelli pagati in Francia, Spagna e Germania. E non si tratta solo di applicare tariffe sociali - così come previsto per esempio nel DPEF - ad alcune fasce di popolazione in sofferenza, ma di attuare una riduzione del costo generalizzata. Il Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea ritiene indispensabile e urgente che in materia di politica energetica siano definiti obiettivi chiari e condivisi con le istituzioni locali e la popolazione e che le linee direttrici debbano fare riferimento a tre questioni: al rispetto del Protocollo di Kyoto (e in questo senso la politica energetica non può essere avocata ad un solo Ministero, ma va concertata con il Ministro dell'ambiente), all'approvazione del Piano energetico nazionale, necessario a individuare le strategie di sviluppo a partire dal fabbisogno reale, ed alla definizione del ruolo italiano in Europa.

Signor Presidente, annuncio la decisione del Gruppo dell'UDC di non partecipare al voto sul disegno di legge che prevede l'abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale. Ciò perché se questa duplice abrogazione di decreti-legge, uno del 2001 del Governo Amato, l'altro del 2005 del Governo Berlusconi, è resa necessaria al fine di evitare le pesanti sanzioni europee che attenderebbero l'Italia ove non si adeguasse alla sentenza del 2 giugno 2005 della Corte di giustizia europea, evidenziato che il nostro Paese vive una schizofrenia tra la situazione interna (che riguarda, per esempio, i costi che le famiglie e le aziende sopportano per acquistare energia e tariffe troppo alte e doppie rispetto a concorrenti Paesi europei) e il contesto continentale, dove in tema di privatizzazione del settore dell'energia elettrica non abbiamo da prendere lezioni da nessuno, essendo stati zelanti persino nella stessa missione della Commissione europea. Se, da un lato, la privatizzazione non ha avuto un effetto diretto sulla riduzione delle tariffe, almeno nell'immediato, dall'altro, ci vede con un passo più svelto rispetto ad altri Paesi europei, che su questo cammino sono più indietro di noi e sono oggetto di messa in mora da parte della stessa Unione Europea. Questa schizofrenia, e vengo al motivo per il quale l'UDC non parteciperà al voto, è aggravata dall'inerzia che sembra soffocare la politica del Governo Prodi in questo ambito. In particolare, vale la pena ricordare che le norme che sono oggetto di questa proposta di abrogazione sono note per garantire non un anacronistico protezionismo nazionale nei confronti dei francesi, quanto condizioni di reciprocità che assicurino al nostro Paese di non perdere competitività sul mercato europeo, per il solo fatto di essere stati zelanti nel cammino delle privatizzazioni. È successo infatti che l'EDF, che Oltralpe è sostanzialmente monopolista dell'energia, abbia acquistato partecipazioni di notevole entità nell'italiana Edison Spa, sfruttando, va detto, la posizione di comodo di cui EDF gode nel suo Paese. Può sfruttare infatti le risorse finanziarie che le vengono dalla rendita monopolista e, non avendo azionariato privato, non ha obblighi di distribuzione di dividendi tra gli azionisti. È stato questo il motivo di quei due provvedimenti legislativi che si vogliono oggi abrogare: assicurare il rispetto di un accordo bilaterale Italia-Francia volto a favorire l'ingresso di nuove società nel mercato dell'energia francese. Qual è stato il risultato e qual è il rischio che corriamo se saremo costretti a patire l'inerzia del Governo? Abbiamo visto cosa è successo quando venne tentata l'OPA su Suez: la Francia si è messa in mezzo per il tramite di *Gaz de France* facendo fallire l'acquisto. Per converso, abrogando le norme in parola, consentiremo alla Francia di dispiegare tutta la forza azionaria che le viene dalle quote di partecipazione nella società. Per questo, signor Presidente, la nostra non partecipazione al voto sta lì, responsabilmente a sottolineare che non staremo a guardare mentre il Governo lascerà che il Paese perda in competitività senza alcuna garanzia di reciprocità. Non staremo a guardare mentre il presidente Prodi, distratto da qualche provvedimento di facciata in tema di liberalizzazioni, lascerà che l'Italia venga colonizzata da società estere senza almeno garanzie in ordine alle necessarie condizioni di pari opportunità mercantilistiche per le nostre aziende. aziende. Da questo deriverà infatti un ulteriore danno per le famiglie e per il tessuto produttivo in Italia. Il ricordo dei *black out* di due anni fa o la crisi che lo scorso inverno abbiamo vissuto a proposito dell'approvvigionamento del gas è ancora troppo vivo perché si possa fare a meno di tener presente che l'interesse del nostro Paese va oltre il semplice smarcarsi dal rischio di pagare una sanzione. Queste sono le motivazioni che ci spingono a non partecipare al voto, evidenziando un'astensione che non vuole essere considerata un voto contrario, ma in questo caso è e vuole essere tecnicamente un'astensione politica.

Signor Presidente, debbo dire che trovo singolare la dichiarazione dell'onorevole senatore Maninetti rispetto alla non partecipazione al voto che al Senato equivale, al di là dell'arrampicamento sui vetri, ad un voto contrario; atteggiamento diverso da quello tenuto diverso da quello tenuto dal suo Gruppo in Commissione e alla Camera. Siamo di fronte ad un provvedimento dalla portata molto limitata, come veniva ricordato dal relatore e dall'intervento nel dibattito della senatrice Alfonzi, che è praticamente un atto dovuto. Sarebbe inerte il Governo se non prendesse un provvedimento di fronte al fatto che due provvedimenti di due Governi di colore diverso, il Governo Amato con il provvedimento detto Enrico Letta e il provvedimento del Governo Berlusconi del 2005, sono entrambi incappati nella sanzione della Corte di giustizia europea per una sorta di *par condicio*, come ironicamente potremmo dire. Di fronte a questa situazione, è evidente che qualunque misura che tendesse, come quella del 2005, ad annacquare il divieto di presenza nel voto elevando la quota del 2 per cento non risolverebbe le obiezioni che ci provengono dall'Europa. Quindi, non possiamo fare altro, a meno di non incappare in sanzioni pecuniarie che ricadrebbero sulle spalle dei cittadini italiani, che assumere una misura di cancellazione della norma del 2001 del Governo Amato e della norma del 2005 del Governo Berlusconi; *par condicio*, come vedete. Non è vero che nel frattempo il Governo è privo di difese di fronte ad eventuali scalate di colossi energetici con prevalenza di partecipazione pubblica che vengono da altri Paesi europei perché rimane in vita la norma della cosiddetta Marzano II, cioè il comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 39 del 2004, che dà il potere, qualora il Governo lo ravvisi, entro trenta giorni, di intervenire se un campione nazionale è in pericolo. È un potere non automatico, ma è una deterrenza che serve per bloccare intenzioni di conquista rapida e priva di condizionamenti da parte di monopoli pubblici o privati esterni al nostro Paese. Inoltre, il senatore Maninetti e le forze di opposizione sanno che il Governo è talmente poco inerte che già presso questo ramo del Parlamento giace - ed è pronto alla discussione - un disegno di legge più generale sul problema della liberalizzazione nel campo energetico e del potenziamento della produzione di energia con fonti rinnovabile che costituisce un tassello essenziale anche per far fronte a quelle possibili emergenze rispetto alle quali questo Governo è già attivato sotto il profilo amministrativo, cioè quelle che vogliono evitare un *black out* di berlusconiana memoria. come avvenne in passato. La discussione generale sugli indirizzi della politica energetica del nostro Governo e del nostro Paese nel contesto internazionale è quindi assicurata e già incardinata in questo ramo del Parlamento e sarebbe improprio

illustrato dalla senatrice Alfonzi, che richiama il Governo ad un impegno ancor più generale, ossia l'elaborazione di un piano energetico nazionale, tramite anche una Conferenza nazionale sull'energia che valuti il fabbisogno effettivo e quanto può essere prodotto, affinché vi sia anche una partecipazione italiana sul mercato internazionale. Nel provvedimento in esame vi è l'immediatezza, l'emergenza, il collegamento al quadro giù generale, una clausola di salvaguardia da scalate provenienti da altri colossi energetici,

Presidente, prendiamo atto che il provvedimento in esame si conforma ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che impone all'Italia l'abrogazione delle leggi n. 301 del 2001 n. 131 del 2005, pena consistenti sanzioni. Ciò non toglie che il Governo avrebbe potuto e dovuto illustrare meglio in Commissione i suoi intendimenti sulla materia e, in particolare, sulla questione della reciprocità, che al momento manca in altri Stati quali, ad esempio, la Francia. Su tali aspetti di vitale importanza ignoriamo le posizioni del Governo, che peraltro, dai continui voti di fiducia che richiede, dimostra insufficiente energia per il proprio funzionamento e per la propria credibilità.

siano tali da convincere dell'opportunità e della necessità di approvare questo provvedimento, che - lo voglio ricordare

proiezioni verso la costruzione del piano energetico nazionale, con tutte le attenzioni e le indicazioni contenute nell'ordine del giorno G1, che il Governo ha recepito, siano tali da rispondere anche ad una legittima interlocuzione e ad una legittima domanda che gli interventi dell'opposizione hanno proposto. *(Applausi Signor Presidente, colleghi, comprendiamo tutti le ragioni sottostanti a questo provvedimento di legge. Si tratta di recepire una sentenza della Corte di giustizia europea e di rispondere ad una richiesta precisa della Commissione europea. Ciò detto e ciò riconosciuto, va tuttavia sottolineato che non è vero, sottosegretario Gianni, che nel disegno di legge depositato presso questa Camera riguardante le problematiche dell'energia vi siano accenni o precisazioni riguardo alle tematiche di grandissimo peso (la reciprocità, la liberalizzazione dei mercati), sottostanti al problema

astensione dal voto per quanto riguarda Forza Italia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento ha avuto in Commissione un voto unanime. Prendiamo ora atto che nel corso del dibattito in Aula c'è stata una serie di differenziazioni.

La prima è che, a mio avviso, si rende assolutamente necessario giungere rapidamente all'abrogazione dei due provvedimenti normativi in tema di partecipazioni in società operanti nel mercato dell'energia elettrica

della Corte di giustizia europea che, con propria sentenza del 6 aprile 2006, ha messo sotto infrazione il nostro Paese. Corriamo pertanto il rischio di dover pagare 250 milioni di euro se non si pone rimedio a questa situazione di carattere legislativo.

Riconosco che forse è irrituale il tipo di richiamo, però vorrei pregare i colleghi - ovviamente è legittima ogni posizione - di non attribuire ad altri voti che non hanno espresso. espresso. Mi sono informato, non essendo membro della Commissione, dai colleghi del mio Gruppo parlamentare, in quanto ero rimasto colpito dalle tesi che sostengono che questo provvedimento è stato approvato all'unanimità. Non è stato approvato all'unanimità alla Camera, non è stato approvato all'unanimità nemmeno in Commissione al Senato. Bisogna avere quindi l'onestà di dire che, nella seduta del 26 luglio, questo provvedimento è passato a maggioranza, come risulta dal resoconto del Senato; non si può falsamente sostenere che è stato votato all'unanimità.

Colleghi, poiché mi sembra una questione su cui c'è la possibilità di una verifica, mi rimetterò solo agli atti scritti delle Commissioni. Non facciamo una Commissione d'inchiesta per una cosa del genere!

riguarda l'autorizzazione fantasma a porre la fiducia sul decreto-legge Bersani-Visco.

perché il comunicato stampa ha omesso - cosa che di solito non avviene - di includere questo importantissimo atto del Consiglio dei ministri, se è avvenuto. Ebbene, nel video della conferenza stampa il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nonché segretario del Consiglio dei ministri (com'è precisato nel nel comunicato stampa), alla domanda precisa se l'autorizzazione ad apporre la fiducia (senza la decisione che per forza questa autorizzazione andasse usata) si riferisse

del Senato sicuramente hanno trasmesso saranno ascoltate, in modo che io possa ricevere la risposta del Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana.